La seduta è aperta

brevemente, cogliendo l'occasione della presenza del Ministro dell'interno. Il nostro Paese ha svolto una meritoria opera di sostegno per ottenere un voto dell'ONU per la moratoria sulla pena di morte. nei giorni scorsi ho visitato il quartiere San Giovanni di Napoli e mi chiedo perché, con l'autorizzazione a realizzare un impianto a turbogas, si sia deciso di applicare la pena di morte ad un imprecisato numero di abitanti di quella città, città, senza nemmeno applicare una parvenza di tutela della salute rappresentata dalle procedure obbligatorie di valutazione di impatto ambientale. Sono lavori illegittimi e in violazione ad ogni elementare regola di tutela della salute dei cittadini. stesso avviene a Modugno, dove gli stessi enti locali rinunciano a verificare l'osservanza delle pur labili disposizioni da essi emanate. Quello dei turbogas è un *business* osceno, che l'Organizzazione mondiale della sanità, pur fermandosi alle PM10 (e quindi non calcolando il devastante impatto delle nanopolveri) stabilisce portatore di morti, malattie invalidanti e danni permanenti al sistema cardiovascolare, alle vie respiratorie ed all'apparato digerente. Ho già presentato, in data 16 maggio, l'interrogazione

PRESIDENTE. Senatore Rossi, sarà nostra cura sollecitare le interrogazioni a cui lei ha fatto riferimento. suo tramite alla seconda carica dello Stato, perché mi auguro voglia far sentire la sua autorevole voce. Non vorrei che, a causa delle protezioni politiche delle numerose società coinvolte nel grande affare delle turbogas,

che oggi il Consiglio di Stato ha dato torto al ministro dell'economia Tommaso Padoa Schioppa in merito al suo ricorso contro la sentenza che ha reintegrato il consigliere di amministrazione RAI Angelo Maria Petroni, illegittimamente estromesso dal Governo e dal Ministro dell'economia*. (Applausi dal quel Ministro, che oggi si vede dire dal Consiglio di Stato che la sua è una paccottiglia propagandistica, ha preso in giro il Parlamento, sostenendo dati e notizie false in ordine allo stato di salute dell'azienda sul piano economico, degli ascolti e della sua organizzazione interna, e ha proceduto ad un atto che oggi risulta essere ampiamente illegittimo, come dicono gli organi giurisdizionali di questo Paese, sarebbe il caso, signor Presidente, che quel Ministro tornasse per cospargersi il capo di guano, dopo averlo cosparso sulle istituzioni del Paese. Mi auguro, pertanto, che sia al più presto convocato in quest'Aula. *(Applausi

che sono parte integrante dell'Unione nazionale combattenti e reduci, ente morale. Sta avvenendo qualcosa che passa sotto silenzio. Questi vigilanti si trovano in una condizione molto grave, dovuta a una situazione debitoria dell'ente morale.

di vigilanza Urbe» è entrato un po' nella storia dei cittadini romani, non tanto dal 1934, quando esso fu costituito, ma con un film, «Un americano a Roma», che parla del vigilante in bicicletta che va a verificare

Nei prossimi giorni è stata data assicurazione che questi sindacati saranno chiamati a un tavolo tecnico.

per quanto potrà accadere nei prossimi giorni.

perché le inefficienze di un sistema provocano sempre la nascita di anticorpi, che non sempre risultano benefici. Se questo principio, Presidente, volessimo poi applicarlo a ciò che sta accadendo oggi sulla riforma della legge elettorale, ne ricaveremmo la triste conclusione che le istituzioni non esistono più e che pertanto la supplenza esterna deve essere accettata purtroppo come un effetto fisiologico. Presidente, sarò ancora più chiaro. Un uomo chiamato Walter, che pur non sedendo in Parlamento pensa di essere l'imperatore di una Roma d'altri tempi, ha deciso di sostituirsi alle istituzioni e, dall'esterno, ha unilateralmente scelto di dettare i tempi e di decidere il merito delle questioni che poi il Parlamento dovrà limitarsi a ratificare. Egli ha incontrato i Presidenti delle Assemblee, ha visto le delegazioni dei partiti, ha informato nottetempo il Governo e ha deciso la linea che comunicherà

sospese, i vertici di Camera e Senato sono stati spogliati di ogni prerogativa di coordinamento dell'azione istituzionale ed il Governo è stato privato di ogni possibilità di mediazione. Insomma, le istituzioni sono state svuotate e saccheggiate in nome di un plebiscitarismo fasullo che in Italia non ha mai prodotto nulla di buono. La sovranità del Parlamento è stata violata proprio rispetto alla sua più alta funzione, quella legislativa, e rispetto alla materia più delicata e sensibile, quella elettorale.

è la sovranità popolare che viene sospesa. Illustri colleghi, ritengo sommessamente che non possiamo continuare così e lei, signor Presidente, che a norma della Costituzione e dell'articolo 8 del nostro Regolamento rappresenta tutti noi,

che ha fornito non corrisponde affatto alla realtà. La Commissione affari costituzionali del Senato - e, quindi, la sede istituzionale (l'Ufficio di Presidenza) - oggi si è riunita e ha lavorato per

che sia la RAI sia il Ministero hanno dovuto pagare non so quanto per assoldare illustri avvocati affinché seguissero le pratiche. Quindi, nel momento in cui il Paese non ha i soldi per le autostrade, chi pagherà le cose inutili?

Signor Presidente, la sentenza odierna del Consiglio di Stato è troppo importante per non attirare l'attenzione del Parlamento e, in questo caso, del Senato. A nome del mio Gruppo, proprio giovedì scorso, quindi qualche giorno fa, avevo pregato il ministro delle comunicazioni Gentiloni di dissociarsi rispetto alla politica proterva e arrogante assunta, fino a quel momento, dal ministro Padoa-Schioppa, relativamente alla questione Il ministro Gentiloni, invece, ha ritenuto opportuno proseguire su tale strada e solidarizzare con il ministro Padoa-Schioppa. Anche il Gruppo di Alleanza Nazionale si associa a quanto dicevano i colleghi: è indispensabile che il ministro delle comunicazioni Gentiloni ed il ministro dell'economia Padoa-Schioppa vengano in Aula a riferire sullo stato attuale - ma soprattutto futuro - della RAI.

Presidente, intervengo sull'argomento, per far mie, anche a nome della componente del movimento politico La Destra, le affermazioni dei colleghi Galli e Butti. Credo che il Senato non possa non chiedere, nella sua globalità, un nuovo dibattito sulla questione RAI. Ma le dico di più, signor Presidente. Credo che la Presidenza del Senato debba muovere dei passi nei confronti del Ministro dell'economia per alcune elementari ragioni. In quest'Aula c'è stato un dibattito molto acceso, con tantissime votazioni che non hanno sortito alcun effetto. Il Ministro dell'economia è stato convocato, con delibera dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, dall'organismo bicamerale per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - la Commissione Landolfi - e si è ben guardato dall'adempiere ad un dovere costituzionale: è la Costituzione, sono i Regolamenti parlamentari a prevedere che il Governo, se richiesto, ha l'obbligo di partecipare alle sedute.

Ebbene, signor Presidente, il ministro Padoa-Schioppa, con la rimozione (illecita: oggi lo possiamo dire) del consigliere Petroni, ha perso sia al TAR che al Consiglio di Stato. Un Ministro che colleziona queste brutte figure dimostra di non conoscere la legge e di non essere adatto al ruolo che ricopre. Per questo solleciterei i colleghi della Casa delle Libertà (se possiamo ancora chiamarla così) a prevedere la presentazione di una mozione di sfiducia individuale. Ma in questo momento credo ci sia necessità di ottenere chiarezza in quest'Aula e prego la Presidenza del Senato di adoperarsi con i suoi buoni uffici affinché la nostra richiesta possa essere esaudita, perché è inaccettabile che la Rai versi ancora in queste condizioni. Signor Presidente, la notizia che abbiamo ricevuto è di straordinaria gravità. In questa vicenda il Governo ha mostrato un forte disprezzo per il Parlamento, per la Camera e per il Senato. Ammonito in Commissione di vigilanza dei sul fatto che il referente del consiglio di amministrazione è la Commissione di vigilanza medesima e non, autonomamente, il Ministro dell'economia,

per analogia, una norma che gli consentiva di procedere alla sostituzione del consigliere Petroni sulla base del codice civile, quando è noto a tutti che esiste una legge specifica che vincola le nomine del consiglio di amministrazione della Rai ad una procedura complessa, il cui punto di riferimento essenziale è il Parlamento e quindi la Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale - come ha detto una volta la Corte costituzionale - è il vero azionista di riferimento.

Abbiamo chiesto ai Presidenti della Camera e del Senato, con lettera del presidente della Commissione di vigilanza, di sollevare una questione costituzionale di conflitto di competenze e il Ministro dell'economia non ne ha voluto tenere Non si tratta di un incidente di percorso, ma della stigmatizzazione, da parte della magistratura amministrativa, di un comportamento gravemente lesivo delle prerogative del Parlamento. Il Ministro dell'economia (ma anche il Ministro delle comunicazioni)

delle valutazioni che qui sono state espresse da più di un Gruppo, rispetto alla necessità di valutare le forme con le quali si può porre in essere un dibattito sulle ultime vicende riguardanti il Consiglio d'amministrazione della RAI. Devo dire al senatore Manzione che dire al senatore Manzione che la Presidenza del Senato non può che apprezzare le valutazioni che tendono a riportare nell'alveo legittimo e legittimato, cioè il Parlamento, in questo caso il Senato, una discussione delicata ed importante come quella dei sistemi elettorali, di cui liberamente il Parlamento doterà il Paese. Va da sè che nessuno può impedire il libero dibattito politico. L'aspetto fondamentale mi sembra l'abbia sottolineato il Presidente della 1a Commissione: la prossima settimana inizierà, con le modalità previste dal Regolamento e dal lavoro della Commissione, il dibattito sui disegni di

Signor Presidente, signor Ministro, nella

data l'importanza e la complessità del problema che investe un settore molto delicato dei rapporti del nostro Paese con il resto della Comunità.

modo precipuo allo spirito comunitario che vorrebbe una Europa spazio di libertà, giustizia e sicurezza - ricordiamo il *summit* di Tampere nel 1999 all'interno del quale nessuno di questi tre valori fosse assunto come prevalente sugli altri, dato che appunto non vi è un ordine di priorità ma sola una esigenza imperativa di armonizzazione degli stessi, mentre ci sembra che il fattore sicurezza sempre più vada assumendo caratteri assorbenti e prevalenti. Le limitazioni al diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione andrebbero innanzitutto specificate - in merito ci auguriamo che alcuni nostri emendamenti vengano accolti e che in questo senso si determini anche il Governo

dato che dalla violazione di norme comportamentali, come quelle indicate dal decreto, deriva una sanzione altamente afflittiva, quale l'espulsione. Vorremmo, cioè, che non ci fosse un criterio vago di interpretazione, ma che la pericolosità che la pericolosità fosse attuale e non riferibile magari ad altre espulsioni o ad altre violazioni di legge commesse nel passato chissà dove e chissà quando. Contemporaneamente andrebbe stabilito che il potere del Ministro dell'interno e dei prefetti - un potere discrezionale - fosse sottoposto ad un giudizio e ad un controllo giurisdizionale di un giudice monocratico ordinario, dovendo quest'ultimo confrontarsi con una normazione tassativa per fattispecie e non con la discrezionalità amministrativa; un giudice ordinario che istituzionalmente è abituato a confrontarsi con le norme e non, come i giudici amministrativi, con la discrezionalità. Va infine rispettata la dignità delle persone che si trovano sul territorio nazionale, siano esse comunitarie o extracomunitarie,

Non vorremmo cioè che questo decreto comportasse delle violazioni di legge che potrebbero anche risultare confliggenti confliggenti con il nostro ruolo all'interno della Comunità Europea, la quale, intesa questa volta come Parlamento europeo, già si è mostrata molto allarmata la piega che stanno prendendo le questioni dell'espulsione nel nostro Paese. Lostesso Parlamento si è già espresso

anche perché, dobbiamo riconoscere, e questo lo hanno sottolineato in molti, che questa urgenza e questa necessità di intervento erano state ritenute insussistenti fino pochi giorni prima poi esplose con l'omicidio della povera signora Reggiani. Credo che un Paese serio non dovrebbe prendere provvedimenti *ad* *horas*, collegati ad un'emergenza.

sembrano poi essere orientati verso i cittadini più poveri dell'Unione Europea, in questo caso verso i rumeni.

quali voglio ricordare che questi nostrifratelli e sorelle comunitari ed extracomunitari avrebbero diritto ad un trattamento più umano. Ricordo - e chiudo - un vecchio *spiritual* dei negri d'America, il quale, letteralmente, dice: "Tutti i figli di Dio hanno le ali". Speriamo che anche il nostro Parlamento si ricordi di questa uguaglianza.

anche morali, nel nostro tessuto economico, istituzionale e di vita quotidiana. Parliamo della sicurezza legata a quei piccoli fatti, che violentano, in maniera simbolica o in modo materiale e diretto, la nostra parte più intima, la nostra casa, la nostra famiglia, il nostro luogo di lavoro,

un lato, egli ritiene che certi fatti possano essere più facilmente controllati rispetto ai grandi fenomeni criminali; dall'altro, nutre una maggiore preoccupazione perché si sente completamente indifeso, pur in presenza di mezzi e modi

ed è anche divenuto un problema popolare, nel senso che riguarda il popolo nella accezione più ampia del termine. Non riguarda più soltanto i ceti agiati Non riguarda più soltanto i ceti agiati o i possessori di redditi e patrimoni elevati, ma colpisce indistintamente tutti i cittadini. Non è un caso che in tutte le città

Questo fatto dovrebbe unire tutte le forze politiche parlamentari, al di là delle posizioni ideologiche, a considerare il problema sicurezza come un problema di tutti.

di voler abbassare la guardia di fronte a fenomeni criminali che provengono soprattutto dagli extracomunitari per lo più entrati clandestinamente. Adesso si evidenzia una novità

verso i quali si è determinata una politica di ingressi e di mancanza di controlli sul territorio che rende ancora più preoccupanti i fenomeni criminali collegati a queste popolazioni. Ministro

questo ritardo nel presentare il pacchetto sicurezza? Evidentemente, perché nel centro-sinistra vi è una frattura tra il permissivismo, il buonismo, il lassismo della sinistra radicale e un maggior senso di responsabilità

a seguito di quell'orribile delitto avvenuto a Roma, una parte di questo pacchetto si traduce in un decreto‑legge.

riemergono quelle sensibilità e quelle ideologie di tutela a tutti i costi di chi è ritenuto,

attraverso i giornali della sinistra, che ha avvelenato il dibattito. La posizione del centro-destra è sempre stata molto chiara: noi riteniamo che il decreto-legge sia intervenuto in ritardo

serietà di questo decreto legge. Signor Presidente, signor Ministro, nella cultura e nel senso comune dei Paesi dell'Europa occidentale la città è tradizionalmente rappresentata come una collettività omogenea, che si specchia in se stessa e che riconosce a se stessa un'identità. Al di là della città c'è il mondo, con le sue diversità, abitato da popolazioni lontane dalle nostre. Questa è la tradizione, ma nel nostro presente il mondo entra nella città. Chi è diverso da noi non è più lontano, fa parte del nostro stesso *vicus*, non sta al di là del fiume, non è un rivale ma un nostro vicino, che vive con noi. La dislocazione delle forze produttive, la forma dei rapporti fra vita e consumi nelle regioni più sviluppate del mondo fanno sì

È un movimento dal Sud verso il Nord, da Est verso Ovest, che non è possibile fermare o ricacciare indietro: dobbiamo governarlo

La ringrazio, Presidente. Dobbiamo governarlo in modo che le persone che vengono da altri Paesi, e vengono qui per stare con noi, rispettino le leggi dello Stato che li ospita. Le tensioni riguardanti i migranti che provengono da Paesi esterni all'Unione non sono l'unico problema Senatore Mazzarello, sta disturbando il suo collega. appartenenti agli Stati membri dell'Unione. È vero, in questi ultimi mesi, da più parti è stato segnalato un problema specifico - che faremmo male ad ignorare - legato all'ingresso di un alto numero di persone, provenienti dalla Romania, Stato membro dell'Unione Europea, nel nostro Paese. Segnaliamo questo problema poiché accanto a lavoratori, a persone oneste, che vengono qui e che vivono accanto a noi, spesso in condizioni assai disagiate, vi sono anche gruppi criminali che si sono insediati in Lombardia e a Roma, e che sono dediti al traffico della droga e, in particolare, per quello che abbiamo saputo nei mesi scorsi, dell'eroina. Dobbiamo contrastare questi gruppi criminali, dobbiamo governare le tensioni, cercando progressivamente di attenuarle e di fare in modo che le persone diverse da noi, che vivono con noi, diventino sempre più vicine e sempre meno rivali, sempre più parte della nostra collettività e sempre meno ostili o non integrate. Sbaglia chi pensa oggi di governare l'Italia, ed in particolare

che spesso la paura nelle nostre società, nella vita quotidiana delle nostre città è un dato reale, esiste. Vi è la percezione di un pericolo strisciante, diffuso stato d'animo di insicurezza nei ceti popolari. Credo sia giusto che un Governo di orientamento democratico, che tra le sue idee guida ha anche l'idea di uguaglianza - uguaglianza nel rispetto delle leggi e nel modo in cui sono trattate le persone più deboli - si ponga l'obiettivo di dare più sicurezza ai quartieri popolari delle città, alle persone che hanno meno strumenti per difendersi. Le donne scippate, le persone anziane che vengono derubate quando vanno all'ufficio postale per ritirare la pensione; sono loro i più deboli. I negozi rapinati o svaligiati, quelli che non hanno sofisticati sistemi di allarme, appartengono a persone si riferiscono a mondi sociali che hanno meno difese, che sono più esposti. Ebbene, è un dovere dello Stato dare sicurezza a quei ceti popolari, a quelle persone deboli, a quei negozianti. È vero, questo decreto‑legge nasce da un episodio drammatico; io non vedo niente di censurabile nel fatto che di fronte ad un episodio drammatico, che scuote l'opinione pubblica, che rivela l'esistenza di una condizione di tensione e la e la percezione aspra ed ampia di un pericolo, si intervenga con norme urgenti e necessarie, purché tali norme, che apprestano strumenti di tutela e servono a garantire meglio il diritto alla sicurezza, non siano arbitrarie, non siano tali da calpestare i diritti costituzionali e le libertà.

in quest'Aula - i diritti siano salvaguardati, le garanzie siano efficaci e l'esigenza di sicurezza trovi uno strumento in più per essere soddisfatta. Le nuove norme disciplinano quattro tipi di provvedimenti, ciascuno con un fondamento diverso. Sono provvedimenti di allontanamento tutti ai medesimi destinatari, vale a dire ai cittadini dell'Unione, e ai loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, verso i quali sono possibili espulsioni mirate:

nei confronti della circolazione dei cittadini europei entro il territorio dell'Unione. Pur tenendo fermi i principi della direttiva europea, è possibile procedere all'espulsione per motivi di pubblica sicurezza sulla base del decreto-legge che stiamo discutendo, nonché a forme di espulsione immediata, decise dal Prefetto ed attuate dal Questore, per «motivi imperativi di pubblica sicurezza». Quest'ultima formula, che non è presente nel linguaggio dell'ordinamento italiano, viene direttamente ricavata dalla direttiva europea: i «motivi imperativi di pubblica sicurezza» sono motivi particolarmente gravi. Credo che nella discussione di oggi si potrà emendare il testo del decreto, rendendo più stringente il riferimento ai criteri che possono dar luogo all'espulsione per «motivi imperativi di pubblica sicurezza». Vi è anche una nuova disciplina relativa all'allontanamento di persone nei confronti delle quali siano cessate le condizioni che legittimano il diritto al soggiorno.

rimanendo, come dobbiamo, entro i limiti della normativa europea. Credo quindi che nel dibattito di oggi si possano confrontare liberamente le opinioni della maggioranza e dell'opposizione, che vi possa essere un contributo da più parti per arricchire queste norme e per contribuire, in tempi rapidi, alla conversione del decreto-legge, con le modificazioni idonee a rafforzare

Questa è, a mio avviso, un'occasione nella quale, come diceva or ora il senatore Brutti, è francamente possibile che si confrontino esigenze proposte di miglioramento di questo decreto che possano riflettere orientamenti comuni, nei limiti segnati dalla direttiva comunitaria e, prima ancora, dalla Costituzione della Repubblica.

esse facevano parte di un disegno di legge, approvato in precedenza dal Consiglio dei ministri, e sono diventate decreto, certo, dopo la tragica morte della signora Reggiani.

Avete ceduto alle ragioni dell'emotività, si è detto. Ho ritenuto necessario questo decreto perché, dopo quella terribile stavano prendendo piede a Roma, e non soltanto a Roma, delle reazioni xenofobe che investivano la comunità rumena nel suo insieme. Davanti a reazioni di quella natura era importante che ci dotassimo della capacità di una risposta immediata nei confronti dei cittadini comunitari pericolosi per la sicurezza pubblica, allo scopo di aiutare i nostri concittadini a distinguere tra il cittadino non nazionale delinquente e il cittadino non nazionale che non ha nulla della delinquenza. Vorrei che questo fosse tenuto presente. *(Brusìo).* Colleghi,

dobbiamo un grande rispetto al dibattito che si sta svolgendo. Poiché vi è una interlocuzione del Ministro con molti degli intervenuti, pregherei i colleghi, compreso il collega Coronella, di seguire il dibattito stando al loro posto. Il tema è importante e torneranno alcuni degli spunti nelle piccole discussioni in cui ciascuno si accalorerà sul suo emendamento. Vorrei anche spiegare alcune direttrici che ritengo giusto che il Governo segua davanti agli emendamenti. Quindi, ciò non è irrilevante. Il primo punto che vorrei mettere in evidenza è il buon fondamento del decreto nella necessità di distinguere tra i i cittadini comunitari pericolosi per la sicurezza pubblica e gli altri, ad evitare lo scatenamento di onde emotive che finiscono per trattare tutti i non nazionali nella stessa maniera. Isolare e colpire con sollecitudine i pericolosi aiutava a questo scopo; di qui il decreto, il decreto, che naturalmente, proprio per questo (giustamente alcuni di voi lo hanno rilevato), non serviva a essere deportazioni immediate e contestuali di migliaia e migliaia di cittadini comunitari non italiani. Questo è un fatto comunque impensabile in uno Stato di diritto;

Questa è una delle offese più gravi che sono state fatte all'Italia e io, quale rappresentante del Governo italiano, ho dovuto reagire dicendo che non aveva senso. Il decreto è destinato - come prevede la direttiva comunitaria - a colpire, in ragione del loro specifico comportamento, persone che risultino pericolose. Quindi, se lo misurate in base ai numeri, è inutile che vi aspettiate delle cifre da stadio, perché qui non stiamo adunando gli spettatori di una partita, ma isolando dei soggetti pericolosi. Nel giro di un mese, già stati adottati, nell'insieme, oltre 200 provvedimenti. Non amo questa classifica, ma la Francia, che ne ha fatti 775 in un anno, si muove con ritmi analoghi, perché poi il ritmo non mantiene necessariamente le caratteristiche che ha all'inizio. Di questo spero che tutti vogliamo essere consapevoli. Il difetto della direttiva non è quello di non consentirci deportazioni di massa, perché questo non è un difetto. I difetti della direttiva, e ci arriverò rapidamente, sono in realtà altri perché, perché, andando ai singoli punti, vedremo che questa è una direttiva che per taluni specifici aspetti sarebbe bene che il Senato desse un mandato al Governo perché possa, in sede comunitaria, arrivare a modificarla. Ci siamo infatti accorti di aver discusso di norme possibili, utili, che tuttavia si infrangono sui limiti della direttiva e Chi ha visto le carte sulla base delle quali è stato predisposto il giudizio sul decreto del Governo italiano, così come è oggi a Bruxelles, sa che

il decreto, quando lo abbiamo adottato, introducendo le norme del disegno di legge già approvato dal Consiglio dei ministri, serviva, in serviva, in realtà, a precisare e ad articolare meglio le specificità e le modalità per l'espulsione motivata da ragioni di pubblica sicurezza, che il decreto legislativo di attuazione della direttiva adottato a febbraio aveva trattato con una certa sinteticità che finiva per essere limitante. Ricorderete che nel decreto legislativo si era attribuito al solo Ministro il potere di espulsione, finendo così per mettere insieme ragioni di ordine pubblico, ragioni di sicurezza dello Stato e ragioni di sicurezza pubblica, assoggettandole tutte allo stesso trattamento, un trattamento quindi riduttivo. Il cuore della nuova disciplina, e quindi del decreto, era innanzitutto quello di intestare la sicurezza pubblica in via assolutamente prevalente al prefetto, salvo che per i cittadini comunitari già in Italia da più di dieci anni e per i minori; in secondo luogo, di prevedere l'ipotesi distinta dell'espulsione per motivi imperativi di pubblica sicurezza, immediatamente eseguibile dopo la convalida giudiziaria.

davanti - e qui vediamo emergere le difficoltà oggettive della direttiva - in primo luogo, alla difficoltà di definire con certezza la data di ingresso, essenziale per accertare se sono passati i tre mesi a seguito dei quali si deve dimostrare di avere i mezzi di assistenza; in secondo luogo, e ancor di più,

del divieto di reingresso per coloro che sono stati allontanati per motivi diversi dalla sicurezza pubblica e quindi per assenza di mezzi. Venerdì della

e gli ho chiesto: gli allontanati per motivi di insufficienza di mezzi, come li gestite?

ma loro praticano una sorta di rimpatrio assistito, nel senso che danno loro del danaro per invogliarli ad andarsene. Ebbene, gli allontanati ne spendono una parte per il viaggio di andata e ritorno e ritornano la settimana dopo

«I beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante. Lo Stato dovrà esaminare se si tratta di difficoltà temporanee». In sostanza, l'ipotesi è che si sia davanti a singole, limitate, specifiche situazioni

noi dobbiamo modificare la direttiva, per rimuovere l'impossibilità di imporre il divieto di rientro

Ora, che trattamento fare? In assenza di una previsione della direttiva, noi non possiamo espellere dall'Italia sulla base di un'espulsione deliberata in Francia e il mio collega francese è d'accordo con me sul fatto che sarebbe bene che io lo potessi fare, ma io non lo posso fare, perché la direttiva, così com'è congegnata, non attribuisce ai prefetti di ciascun Paese un ruolo di accertamento per l'intero territorio dell'Unione, ma esclusivamente in quanto autorità dello Stato membro da cui l'espulsione avviene. La direttiva può rimuovere questo limite e può configurare il mio prefetto come autorità che adotta un provvedimento riconosciuto nel territorio dell'Unione, ma io, con la mia legislazione nazionale, non posso farlo. Se decido di non farlo - e questo vorrei, colleghi, che fosse chiaro per tutti - non è perché sono assoggettato a un orientamento politico piuttosto che a un altro, ma perché sto rispettando i princìpi della legalità comunitaria, che certe cose mi consente di farle e certe altre non me le permette e sarebbe bene per il prosieguo della nostra discussione che questo principio fosse acquisito da tutti e che fosse la premessa sulla base della quale ci muoviamo

il relatore Sinisi e il presidente Bianco perché, attraverso i lavori della Commissione, è venuto fuori un gran lavoro che permette di migliorare le nostre norme, ma entro i limiti che ho ricordato. Permettetemi, prima di concludere, di fare qualche cenno ai punti che considero importanti e di possibile miglioramento. Circa la questione dell'allontanamento,

come una dichiarazione che ha valenza di ordine e di sicurezza pubblica significa precostituire un fattore presuntivo ai fini della lettura dei comportamenti dell'interessato che la direttiva vieta. Vorrei che i colleghi che avanzano determinate proposte avessero presente sempre l'articolo 27 della direttiva, la quale dichiara che, ai fini dell'espulsione per motivi di sicurezza pubblica «il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave». Di fronte a una direttiva che usa questo linguaccio non posso fare presunzioni e, soprattutto, non posso creare dei ponti surrettizi, in ragione dei quali - mi rivolgo, in particolare, ai giuristi, che qui sono tanti - finisco per trasformare l'allontanamento per mancanza di mezzi in allontanamento per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica. Questo non posso farlo; posso chiedere all'Unione Europea di rafforzare autonomamente l'allontanamento per mancanza di mezzi, ma non posso tirarci il cappello trattando l'uno come se fosse l'altro. Quindi, dare data certa, sì; va bene anche prevedere che vi sia una dichiarazione che la dà, in assenza della quale vi è una presunzione *- iuris* *tantum*, direbbe un giurista - che una prova contraria possa col prevedere che i mezzi di sussistenza debbano essere leciti. Fin da quando è entrata in vigore la direttiva, ho dato disposizioni ai prefetti ed ai questori non tanto di verificare se una persona perbene che guadagna poco raggiunga o superi di dieci euro il livello minimo,

colui che i mezzi di sussistenza li ha, ma difficilmente è in grado di dimostrare che sono leciti. Allora, sottolineare i mezzi leciti è importante e se uno non dimostra di avere mezzi leciti di sussistenza, questi sì che può essere espulso per ragioni di pubblica sicurezza; probabilmente, non per motivi imperativi, ma di pubblica sicurezza perchè poi

che l'allontanamento, con tutti i limiti che presenta finché non è accompagnabile dal divieto di rientro, comporti la cessazione dell'iscrizione anagrafica, perché questo poi implica determinate conseguenze. Per quanto io trovo giusto che si specifichino meglio i motivi imperativi e che si cerchi di conferire alcuni connotati. Noi lo abbiamo fatto in modo generico; il lavoro svolto qui in Parlamento indica motivi più specifici, fa riferimento ai precedenti penali, non in modo tassativo (e questo è giusto e corrisponde anche allo spirito della

(e non sempre ciò viene tenuto presente) e, in quanto operano come ufficiali di Governo, qui e altrove, applicano le leggi della Repubblica, perché gli ufficiali di Governo devono rispettare tutti le leggi della Repubblica.

e che riflette le mie più profonde convinzioni di cittadino e - se volete - di studioso, che, nel 2004, trovai sbagliato, come larghissima parte della dottrina e come lo stesso Consiglio superiore

Giustamente, il Consiglio superiore scrisse, nel suo parere negativo sulla legge del 2004, che "di fronte ai diritti fondamentali di libertà posti in gioco, non può non assumere preminenza l'esigenza di assicurare tutte le garanzie ordinamentali a soggetti che costituiscono, a tutti gli effetti, soggetti deboli e in quest'ottica (...) questi profili possono essere assicurati dalla magistratura professionale". Il giudice di pace era nato per piccole liti civili. Ebbene, nei tardi anni Novanta, una competenza penale che fu prescelta e selezionata in ambiti che non comportassero mai l'erogazione di pene detentive e l'interferenza con la libertà personale. Questo è il quadro normativo in cui si colloca, rispetto al quale avergli affidato la convalida di provvedimenti che attengono alla libertà di persone (siano esse italiane, comunitarie non italiane o non comunitarie) contrasta con un principio cardine del nostro ordinamento. È per questa ragione che noi riteniamo, in questa occasione, come già avevamo proposto di fare nel disegno di legge di riforma della legge sull'immigrazione, che sia attribuito qualunque compito in quest'ambito al giudice di tribunale monocratico. Si possono organizzare turni, non c'è obiezione organizzativa che regga: un tribunale può organizzare turni, assegnare un giudice a questo, e il giudice, nelle 48 ore, lo fa. Io non posso trasferire al ginecologo un'operazione di cardiochirurgia solo perché penso di avere meno cardiochirurghi, soprattutto perché i cardiochirurghi li ho, basta che li sappia organizzare in modo efficiente. Infine, consentitemi di dire una parola brevissima sul problema che è stato sollevato e sul quale voglio tranquillizzare il Senato: la questione della copertura e del come è fatto il bilancio (mi rivolgo anche alla Commissione bilancio). Fra i capitoli di bilancio, oggi, 2007, il 26.24.25, che copre, con 10 milioni, spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica; spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione o respingimento; spese per l'allontanamento dal territorio nazionale di stranieri, a seguito di accordi e convenzioni internazionali. Questo capitolo regge qualunque ipotesi di allontanamento, non presenta problemi giuridici e, una volta tanto, neppure problemi di copertura finanziaria. Vi ringrazio.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, con l'osservazione che i dati contenuti nella relazione tecnica, pur chiarendo l'assenza di problemi di copertura del provvedimento, pongono una questione di rispetto delle regole di costruzione del bilancio secondo il quadro della legislazione vigente». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo, ad eccezione che sulle proposte 1.26, 1.47 e 1.10, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Lei mi scuserà, Presidente, ma essendo l'emendamento arrivato alle ore 16,30, vorrei chiedere alla cortesia del Ministro se poteva indicare quali erano queste strutture destinate per legge, sì da avere un panorama chiaro della situazione.

c'è una sola realtà che propriamente è chiamata di permanenza temporanea ed è quella dei centri di permanenza temporanea; non si comprende la ragione dell'emendamento 1.305 dal momento che già esistono e rientrano nel sistema.

che «i dati contenuti nella relazione tecnica (...) pongono una questione di rispetto delle regole di costruzione del bilancio secondo il quadro della legislazione vigente», ma poi non specifica qual è il problema o la questione che i dati medesimi pongono; poiché non riusciamo a ricavarla per via interpretativa - è un parere molto sintetico - sarebbe interessante capire di che questione si tratta.

con i diritti individuali, in molti enti locali si stanno approvando ordinanze contro gli stranieri che abitano nelle nostre città. Oggi pomeriggio, nel consiglio comunale di Treviso si è discussa, su istanza del sindaco Gobbo, esattamente una di queste ordinanze. Ebbene, vorrei riportare

«Sarebbe giusto fargli capire come ci si comporta usando gli stessi metodi dei nazisti: per ogni trevigiano a cui recano danno o disturbo vengano puniti dieci extracomunitari». Credo che il Parlamento dovrebbe ribellarsi a che nelle nostre istituzioni repubblicane qualcuno possa usare dei termini del genere e rifarsi alle SS, come ha fatto questo consigliere, e credo davvero che il Ministro dell'interno dovrebbe prendere dei provvedimenti, così come dei provvedimenti dovremmo prendere tutti noi per espungere dal nostro Paese dei simili esempi di inciviltà.

in quest'Aula è stato richiamato il partito che mi onoro di rappresentare, mi dica se mi consente di rispondere o meno.

agli occhi di questo sonnolento Palazzo. Mi dispiace che il ministro Amato non sia qui, perché le parole di questo consigliere comunale, il quale è un semplice cittadino che ha a che fare tutti i giorni con quel che accade alla gente comune, che non sta rinchiusa in questa sede o nelle ville o nei Palazzi o nelle *enclave* ben protette a cui sono abituati molti *radical-chic*

a testimoniare il razzismo di cui viene fatto segno troppo spesso il Nord e, in particolare, il Nord-Est. Allora, ben venga una discussione su questo tema.

Signor Presidente, credo sia molto importante capire lo spirito di questo ordine del giorno. Dalle segnalazioni che ci arrivano,

di lavoratori, si prevede un ulteriore aumento delle stesse anche se non commisurate al numero effettivo di richieste pervenuto in precedenza ma ad una astratta e opinabile capacità di assorbimento da parte del tessuto sociale e lavorativo del Paese.

inutile discutere delle modalità di espulsione di poche decine di persone pericolose per l'ordine pubblico quando si dà la possibilità a centinaia di migliaia

un voto favorevole su questo ordine del giorno che impegna il Governo a prendere atto che la situazione del nostro Paese non è compatibile con un allargamento

Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale su questo ordine del giorno, che si inserisce nella scia dell'intervento di replica del ministro Amato. Egli ha richiamato, con dovizia di particolari, alla necessità di attenersi, materia, alle direttive comunitarie, e più in generale, alle linee guide definite in sede europea. Ora, se esiste un insieme di disposizioni, per fortuna non approvate, che si discosta in modo netto dai princìpi europei in materia di immigrazione, è proprio il disegno di legge Ferrero-Amato, che contrasta con uno dei pilastri della politica europea in materia, definito già al Vertice di Siviglia del giugno 2002: quello che stabilisce un collegamento netto

come regola principale, rispetto alla quale una deroga è costituita dall'intimazione o da forme alternative. Come tutti sanno, il disegno di legge Ferrero-Amato stabilisce, in via principale, che l'espulsione sia una sorta di adesione volontaria

confusione introdotto dal disegno di legge circa una corretta disciplina degli arrivi? Infatti, il testo del disegno di legge stabilisce un regime di convenzione con le ONG per disciplinare e selezionare gli ingressi regolari nel nostro Paese, al di fuori di qualsiasi verifica di regolarità prevista dal meccanismo delle ambasciate e dei consolati. dei consolati. In questo ordine del giorno noi non leggiamo un provvedimento contro un altro provvedimento, ma il punto di partenza di una discussione parlamentare seria sul tema dell'immigrazione, che potrebbe snodarsi anche in un confronto tra differenti mozioni. In base all'approfondimento e al voto che il Parlamento

nostro avviso, sufficienti per fissare uno *stop* rispetto a questo disegno di legge e per ripartire su basi razionali.

In questo momento non si tratta di un ordine del giorno qualunque, ma della sostanza della politica sull'immigrazione del Governo della Repubblica. Se questo decreto-legge modifica, nella sostanza, la legge Amato-Ferrero, ne discutiamo e possiamo anche votarlo; se non la modifica, se lo tenga la maggioranza, se lo voti e non ci rompa più le scatole. *(Applausi

del giorno pone semplicemente una questione; invita cioè questo Governo a non modificare le politiche sull'immigrazione del Governo precedente. Mi sembra che, al di là della discussione sulla legge Amato-Ferrero, sia effettivamente un po' troppo e credo che nessuno di noi possa immaginare di dover addirittura sottrarre alcuni settori dalla libera disponibilità legislativa del Governo. Per questa semplicissima ragione, inviteremo i colleghi a votare contro l'ordine del G100.

integrandolo con qualche considerazione che va anche al di là della denuncia che esso contiene, che non può non inquietare tutti coloro che hanno a cuore, non soltanto il dettato delle leggi, ma soprattutto gli effetti che queste leggi hanno sui cittadini, soprattutto sugli inermi, sugli indifesi, sui più deboli, come sono gli immigrati, in particolare quelli clandestini. Già in sede di dibattito generale su questo provvedimento, ho avuto modo di sottolineare come la direttiva 2004/38/CE finisca per essere tradita, manipolata e stiracchiata come un elastico, da ciò che è stato messo a punto dal Governo. Mi spiace doverlo dire, in quanto di questa direttiva fui il relatore - come qualche collega che vedo in Aula ricorderà - durante l'esperienza al Parlamento europeo. Debbo dire che c'è davvero un abisso tra quello che si immagina in un contesto europeo ed in una direttiva, che puntava a dettare termini concreti di accoglienza, prima ancora che di espulsione, e la differenza nel constatare come essa sia stata travisata e, quindi, applicata in maniera distorta. Avevo anche chiesto al ministro Amato di verificare che fine avesse fatto il regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2004; un regolamento che, per la prima volta, assegnava direttamente ai Paesi terzi, di provenienza dei più importanti flussi migratori, ingenti quantitativi di denaro - esattamente 250 milioni di euro all'anno - per provvedere all'origine all'origine di rimediare a questo fenomeno, che come sappiamo non è purtroppo un fenomeno soltanto italiano, ma coinvolge tutti i Paesi membri europei. Questi 250 milioni di euro per cinque anni sarebbero dovuti servire per creare condizioni di accoglienza direttamente nei territori di provenienza, ma soprattutto per promuovere azioni di promozione,

tutti i rischi dell'emigrazione clandestina ed, invece, tutti i vantaggi di forme di emigrazione regolarizzata. Infine, c'è un aspetto che vedo la direttiva 38/2004 è estesa anche a cittadini di Paesi terzi, purché coniugati con cittadini comunitari. Va detto che la direttiva per la prima volta ha esteso - con un voto molto dibattuto e contrastato del Parlamento europeo - la figura di coniuge anche a coloro che fanno parte di unioni di fatto.

torto da una valutazione che non si possa far risalire alla Corte di giustizia, può avviare un ricorso. Quindi, prepariamoci, signor Presidente,

Va detto che la direttiva aveva anche una finalità un po' nascosta, che è stata comunque perseguita, vale a dire quella di limitare o evitare le facili espulsioni

in cui si dovessero espellere realmente i cittadini. Spiace davvero a chi ha partecipato al civilissimo dibattito in Parlamento europeo su questa direttiva

per dare un esempio a tutta l'Europa di come le direttive, pur affidate in maniera molto elastica all'interpretazione dei Paesi membri, potrebbero davvero essere indicatrici di un progresso, di qualche passo avanti. In questo caso, siamo in presenza soltanto del consolidamento di una situazione di criticità che sicuramente non potrà essere risolta dal dettato di questa legge. Quindi siamo a questo ordine del giorno e siamo ancora molto preoccupati per gli effetti che la legge Amato-Ferrero potrà avere non soltanto sul piano nazionale, ma anche per il riflesso di un pessimo esempio da trasferire a livello europeo.

a nome delle forze dell'ordine che hanno manifestato in tutte le piazze d'Italia, gridando il loro senso di impotenza per l'assenza di mezzi, addirittura della benzina con la quale garantire un briciolo di sicurezza ai nostri concittadini! Signor Ministro, le chiedo come sia tollerabile in un Paese civile, dove le forze di polizia si vedono costrette a scendere in piazza, a gridare la loro disperazione perché non possono svolgere il loro lavoro, sentirsi dire: fammi una raccomandazione! Noi, signor Presidente, signor Ministro, non siamo abituati a fare raccomandazioni; noi pretendiamo che questo ordine del giorno sia posto ai voti con il sistema elettronico perché vogliamo far sapere alla Polizia di Stato, ai Carabinieri ed alle polizie locali - che voi ben sapete hanno

Presidente, a sostegno dell'ordine del giorno che reca il suo nome, vorrei far presente all'Assemblea, sperando che anche tra i banchi del centro-sinistra ci sia un po' di attenzione su una questione che incide sulla vita quotidiana alla fine di ciascuno di noi,

che faceva riferimento a benzina ed autovetture delle forze di polizia e a manutenzione delle stesse era pari a 67 milioni di euro. Nella legge finanziaria 2007, i cui effetti continuano a prodursi per qualche giorno ancora, la stessa voce di bilancio (benzina e manutenzione delle autovetture delle forze di polizia) è pari a 27 milioni di euro. Quest'anno le forze di polizia rispetto all'anno precedente hanno avuto 40 milioni di euro in meno su un totale di 67 milioni. di 67 milioni. Ricavo questi dati da una scheda che il Ministro dell'interno qualche mese fa consegnò in Parlamento alla 1a Commissione della Camera nel corso della sua audizione. In quella stessa scheda si segnalava che il 43 per cento delle auto in dotazione alle forze di polizia erano inutilizzate per carenza di manutenzione o di benzina. Si era nel giugno 2007. Quindi ritengo che oggi la situazione sia ancora più grave. Nella finanziaria per il 2008 sono previsti ulteriori tagli. Allora, Presidente, ritengo che il pieno di benzina non sia una questione ideologica e che un ordine del giorno che pone all'attenzione del Governo la necessità, all'interno della legge finanziaria, di riempire finalmente questi serbatoi di carburante per la sicurezza di ciascuno di noi non possa non essere votato dall'intero Senato.

esprimevo l'auspicio che il Governo ascoltasse anche la riflessione dei colleghi della maggioranza su questa materia così delicata. Capisco Capisco pienamente la prudenza e la serietà del Governo, perché comprendo perfettamente che questa materia non si risolve con un ordine del giorno, essendo in questo momento in discussione nell'altro ramo del Parlamento una questione delicata che si chiama legge finanziaria.

confacente e coerente con la preoccupazione degli italiani il tema della sicurezza, credo assuma valore politico nei confronti non solo del Governo ma anche

ringrazio il Governo e, proprio in segno di apertura a tutta l'Aula, quindi sia all'opposizione che alla maggioranza,

in modo chiaro a questo ordine del giorno. Contiamo, per meglio dire speriamo, che poi a questo segua effettivamente uno stanziamento, un impegno reale per dotare le forze dell'ordine dei mezzi necessari, almeno di quelli fondamentali, per espletare il loro servizio, che è pericoloso per coloro che si vi sono impegnati ma che è di grande beneficio per i cittadini; se però questo servizio è addirittura impedito fin dall'inizio dalla dalla mancanza di carburante e dal fatto che i mezzi sono obsoleti è chiaro che ciò non sarebbe possibile. Vorrei ricordare che negli anni della scorsa legislatura si sono dovuti, in più di un'occasione, effettuare dei tagli alla spesa pubblica, ma il settore della sicurezza non è mai stato toccato; nonostante questo, anzi, grazie a questo, in essere un'efficace lotta contro il crimine. In questa legislatura abbiamo assistito ad una serie di tagli. Il collega Mantovano si è soffermato sui tagli alle

sugli stanziamenti destinati alle Forze dell'ordine, cioè a Polizia e Carabinieri, che furono colpiti con tagli di 200 milioni e di 80 milioni di euro per il solo 2006. Un'ulteriore diminuzione è dunque avvenuta con i provvedimenti seguenti;

di assicurare l'esercizio delle funzioni delle forze dell'ordine: non c'è una lira o un centesimo di euro in più. Noi abbiamo presentato, con un emendamento, una proposta di incremento sostanziale del Fondo; ma come può il Ministro dell'interno avere dubbi sul fatto di essere a favore

primo (non vorrei darle il classico bacio della morte) è l'apprezzamento per la sua vena, perché gli ordini del giorno di oggi sono quanto mai puntuali. Il secondo è per il Governo, per avere repentinamente cambiato posizione, peraltro senza motivarla.

In effetti, non che io voglia sminuire il valore letterale dell'ordine del giorno, ma c'è una cosa che dovrebbe apparire ovvia: si chiede di garantire le risorse necessarie alle forze dell'ordine per l'esercizio delle proprie funzioni con riferimento non alle vacanze premio o a chissà cosa, ma al carburante e agli automezzi delle pattuglie: senza questa roba non si fa ordine pubblico. allora, ministro Amato, io apprezzo sinceramente il mutamento di opinione sull'ordine del giorno: prima era una raccomandazione (capisco bene, sottosegretario Lucidi),

che le ha garantito la presentazione di un emendamento alla Camera in legge finanziaria? Oppure è una presa in giro? Perché qui dovrete ritornare con la finanziaria. Ci può garantire il Governo che alla Camera si sta provvedendo per inserire nella legge finanziaria le risorse affinché l'ordine del giorno che stiamo

Colleghi, siamo entrati nel mese di dicembre, il Natale fa diventare tutti più buoni, mi auguro che

parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 13 dicembre. Nel corso di questa settimana, a conclusione dell'esame del decreto-legge in materia di sicurezza, si passerà alla discussione di ratifiche di accordi internazionali e del disegno di legge recante semplificazione di adempimenti sanitari. Nella seduta antimeridiana di giovedì 6 dicembre, ove concluso il decreto-legge sicurezza, inizierà in ogni caso la discussione generale sul disegno di legge collegato concernente i servizi pubblici locali, eventualmente preceduta (in apertura di seduta) da voti su questioni incidentali. Le votazioni degli emendamenti e degli articoli del provvedimento avranno luogo la prossima settimana, a partire dal pomeriggio di martedì 11 dicembre e non oltre la seduta pomeridiana di mercoledì 12. Se possibile, in tali sedute sarà altresì esaminato il decreto-legge recante differimento termini in materia ambientale. L'intera giornata di giovedì 13 sarà dedicata alla discussione generale del disegno di legge relativo al protocollo su lavoro e previdenza. Nel corso della prossima Conferenza dei Capigruppo si procederà alla ripartizione dei tempi per l'esame di tale provvedimento, in quanto collegato alla manovra finanziaria. In ordine al *question time* previsto per le ore 16 di giovedì 6 dicembre, restano confermati gli interventi del Ministro per i rapporti con il Parlamento sui Comune di confine, nonché del ministro Bianchi sui treni pendolari e a lunga percorrenza e sul Gruppo Tirrenia. La questione dell'aeroporto di Vicenza sarà invece oggetto, nel corso della stessa seduta, dell'interrogazione n. 1056, a firma del senatore Ramponi Infine, per quanto concerne i lavori del Senato dei giorni successivi, con particolare riferimento alla terza lettura dei documenti finanziari, la Conferenza dei Capigruppo sarà convocata nella mattinata di giovedì 13 dicembre,

Presidente, vorrei fare questo intervento con grande senso di responsabilità e spero tanto che non possa essere oggetto di fraintendimento da parte di alcuno.

Stiamo esaminando e stiamo entrando nel vivo di un provvedimento delicatissimo, che riguarda la sicurezza dei cittadini italiani. di un provvedimento che conterrà al proprio interno momenti di confronto; non dico di scontro, signor Presidente, perché su questo tema l'opposizione è stata estremamente responsabile: ha votato in Commissione i presupposti di costituzionalità e di urgenza ed ha presentato pochi emendamenti. Ci siamo impegnati affinché quest'Aula esiti definitivamente il testo nella giornata di domani, quindi, così come abbiamo fatto in altre occasioni, non verrà da noi alcun gesto che possa essere individuato o interpretato come ostruzionistico. Proprio per questo clima che abbiamo sempre garantito, e che ci auguriamo di continuare a garantire, e per questa divisione su numeri

Quante volte quest'Aula ha visto approvare o non approvare dei testi anche con votazioni dove i numeri erano pari, a seconda se si trattava o meno di un testo, di un emendamento della maggioranza o dell'opposizione?

Ci rendiamo conto che vi sono degli impegni istituzionali ai quali non vorremmo mai che il Presidente si debba sottrarre, ma vi è anche un calendario dei lavori che già ipotizzava che oggi e domani saremmo stati chiamati a discutere di questo argomento. Credo però che

Presidente Schifani, i turni di Presidenza viaggiano sull'ordine della casualità; quindi, sono d'accordo. Io stesso, in Conferenza dei Capigruppo, per superare il problema (che si pone ora per la maggioranza ora per l'opposizione), ho proposto o che i Vice Presidenti non votino, alla stregua del Presidente, o viceversa che il Vice Presidente che presiede possa votare,

la relazione tecnica per capire il senso di quelle righe, certo non molto numerose, che abbiamo scritto, condensando il nostro parere.

modo conservato l'entità delle risorse presenti nelle unità previsionali di base precedenti; quindi, adesso che dobbiamo provvedere all'allontanamento di un certo numero

all'interno dell'unità previsionale di base, distinguere la quota di risorse destinata all'allontanamento dei cittadini comunitari da quella destinata all'allontanamento dei cittadini non comunitari.

la spiegazione è questa. La relazione tecnica presentata dal Governo con la regolare bollinatura dalla Ragioneria attesta che il parere della Commissione bilancio ha fondamento esattamente nelle cifre che ho cercato di richiamare.

che prevedono che i redditi del cittadino comunitario debbano provenire da fonti lecite e dimostrabili, il che è però stato

sono il frutto di un'attenta riflessione sui contenuti della direttiva e sui princìpi accolti anche nella nostra legislazione interna, interna, che non possono discostarsi da alcuni elementi. Il primo è che fino a tre mesi di soggiorno al cittadino comunitario non può essere richiesto

di iscriversi nella nostra anagrafe, indicando, tra l'altro, anche la dimora, come già prevede il decreto legislativo oggi vigente. L'emendamento che nel caso in cui il cittadino non abbia chiesto l'iscrizione entro i 10 giorni, la sua mancata iscrizione,

perché a questa conoscenza sono collegate situazioni, ragioni sostanzialmente di pubblica sicurezza, in quanto è interesse di pubblica sicurezza sapere dove abitano i propri cittadini? è quest'ultima, perché ragioni di pubblica sicurezza valgono per i cittadini e non possono valere per i cittadini comunitari? Per quale ragione si chiede la registrazione a chi è ospitato in un albergo o a chi chiede ospitalità in un *camping*? Perché abbiamo delle *pruderie* voyeuristiche da soddisfare o perché ragioni di pubblica sicurezza richiedono che chiunque (cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari) alloggi in strutture del genere debba registrarsi, affinché sia consentito un controllo di pubblica sicurezza sulla permanenza sul territorio italiano? Aggiungo, ministro Amato: per quale ragione, all'indomani dell'assassinio di Aldo Moro fu approvato un decreto-legge, tuttora vigente, che fa obbligo a chiunque consegni le chiavi di un fabbricato, in qualsiasi cosa consista questo fabbricato (lo consegni a titolo di vendita, donazione, locazione o addirittura prestito gratuito), di comunicare entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza i dati del consegnatario, dell'acquirente, dell'inquilino, con gli estremi del documento d'identità, pena una salata multa, una salata sanzione di carattere penale e di natura contravvenzionale? È per effettuare rilievi statistici o per motivi di pubblica sicurezza? Allora, perché non possiamo prevedere che la mancata iscrizione, prevista dalla legge di attuazione della direttiva, nelle nostre anagrafi, nel caso sia carente, sia motivo di mancata tutela della pubblica sicurezza e quindi possa dar luogo all'allontanamento immediato? Mi aspetto una risposta dal Ministro. all'osservazione del Ministro, che faceva riferimento alla presunzione prevista nel comma 3 dell'emendamento 1.27, in cui si presume che il cittadino dell'Unione che non abbia fatto questa dichiarazione sia entrato nel nostro territorio tre mesi prima della verifica di questo fatto, che comunque si tratta di una presunzione semplice perché resta salva la prova contraria. Quindi, il combinato disposto di queste due norme dovrebbe consentire una maggiore salvaguardia delle ragioni di ordine pubblico. Invece, l'emendamento del Governo, che sembra porre a carico del cittadino comunitario un obbligo analogo, è in realtà semplicemente la classica foglia di fico perché non costituisce un obbligo ma prevede solo la possibilità per il cittadino comunitario di registrarsi al momento dell'ingresso e comunque non collega a questa mancata registrazione nessuna ragione di tutela della pubblica sicurezza, non cambia nulla sul terreno del provvedimento che si possa adottare.

chiamato il Presidente del Consiglio delle grotte, perché ancora oggi, signor Ministro e colleghi, la residenza in Italia deve essere concessa anche se si vive in una grotta, in una *roulotte* o altro. Lei allora, signor Ministro, aveva detto che qualunque requisito noi avessimo anteposto alla concessione della residenzaci avrebbe assimilato alle dittature di sinistra e di destra,

come del resto è richiesto per il ricongiungimento familiare. Stranamente in Italia si deve concedere la prima residenza in qualsiasi luogo, mentre per il ricongiungimento familiare occorre che la casa sia a norma. Orase il nostro ordinamento si basa sulla prima

che scelgono di venire da noi in modo regolare, di cercarsi un lavoro, di rispettare le nostre leggi e le nostre tradizioni, credo sia un dovere civile garantire, insieme alla residenza, un'abitazione in sintonia con il futuro diritto che avranno di essere cittadini italiani.

Vorrei, se il Presidente ritiene che questo sia il momento adatto, parlare in dichiarazione di voto contro questo emendamento,

Sull'emendamento 1.27. Dicevo, comprendo l'intenzione che ha spinto i colleghi a presentare questo emendamento, ma penso anche che questa esigenza possa essere meglio e più correttamente garantita dall'emendamento del Governo che viene subito dopo,

al nostro esame è quello di dare data certa all'ingresso per non consentire alla persona eventualmente fermata

a quella illustrata dal senatore Pastore il quale, se non ho capito male, fa riferimento all'iscrizione all'anagrafe. Mi permetto sommessamente di osservare che tale iscrizione non ha finalità di pubblica sicurezza. Tra la finalità di pubblica sicurezza e lo sfizio dello Stato di iscrivere la gente in qualche registro,

lo ripeto, vuole tenere distinto il canale dell'espulsione per ragioni di pubblica sicurezza da quello dell'allontanamento per violazione degli obblighi legati alla pura presenza sul territorio. Se uno di questi obblighi lo connetto alle ragioni di pubblica sicurezza unifico i canali che la direttiva chiede al nostro

In relazione a ciò si prevede che la violazione degli obblighi che mi portano all'allontanamento ha l'effetto di cancellare l'iscrizione anagrafica (emendamento 1.301), con le conseguenze che ciò comporta ma non altre. Inoltre, non ha bisogno di essere illustrato l'emendamento

le più diffuse considerazioni hanno indotto, noi del Gruppo parlamentare dell'UDC, a presentare un emendamento per cercare di dare sostanza, oltre che linea politica, alle nostre azioni. Abbiamo evidenziato un atteggiamento del Governo che intende, in qualche modo, dare risposte di politica generale e di concordare su alcuni aspetti, affinché la sicurezza del nostro Paese diventi una priorità, in questo momento storico, anche grazie alle opposizioni, che hanno voluto mettere al centro dell'agenda politica la questione della sicurezza delle nostre famiglie, delle nostre imprese e del nostro Paese in generale. Ci siamo resi conto, signor Ministro, che tutto questo non basta perché, al di là dell'attività legislativa, abbiamo bisogno di passare dalla poesia alla prosa nel tentativo di dare sostanza alle nostre determinazioni politiche. Quindi, il nostro emendamento è in questo spirito.

che il Ministero dell'interno, le Forze dell'ordine, i nostri prefetti hanno bisogno di sinergia ma, soprattutto, di sostanza e di un fondo economicamente all'altezza dell'operazione politica che stiamo svolgendo in questo momento nel nostro Paese.

Noi dell'UDC riteniamo priorità economica che un fondo speciale a disposizione del Ministro dell'interno e, quindi, delle prefetture e delle forze dell'ordine per mezzi e strutture sia finanziato in una misura adeguata. Abbiamo individuato 500 milioni di euro come primo passaggio importante per riuscire a dare forza alle determinazioni politiche, sulle quali possiamo essere tutti d'accordo. Concludo, signor Ministro, dicendo che tutto quello che possiamo fare per trovare in quest'Aula sinergie politiche, lo possiamo fare sui fatti, sulle questioni concrete. Se lei questa sera darà un messaggio di disponibilità a far sì che le politiche sulla sicurezza non siano soltanto un esercizio che riguarda la maggioranza, ma siano patrimonio di tutto il Paese e, quindi, di tutto il Parlamento, noi siamo disposti a dare una mano

del crimine, ma soprattutto al rafforzamento delle nostre prefetture e, dal punto di vista economico e sostanziale, delle forze dell'ordine. *(Applausi dal Gruppo* Signor Presidente, illustro sinteticamente l'emendamento 1.208 che descrive i sistemi e i metodi di ricorso contro i provvedimenti di allontanamento. fa riferimento a sollecitazioni arrivate da diversificate parti politiche, prevedendo, in sintesi, che nei confronti dei provvedimenti dei quali tratta il presente decreto-legge si possa fare ricorso in ogni caso davanti al tribunale in composizione monocratica. L'articolo 22 del decreto-legge legislativo n. 30 del 2007 concerne essenzialmente la questione dell'autorità competente a decidere sul ricorso, e tale articolo, così come proposto in modifica dall'emendamento 1.208, concerne anche i tempi del ricorso, che vengono notevolmente abbreviati

riguardava essenzialmente la definizione del ricorso presentato all'autorità competente e, quindi, il fatto che, nei termini indicati di dieci giorni, il tribunale non si fosse pronunciato. In tal caso, veniva scritto, il ricorso si intendeva accolto; tale punto, che prospetta alcune problematiche particolarmente delicate, è stato estrapolato,

Presidente, l'emendamento 1.300/4 intende rendere obbligatoria e non solo facoltativa la dichiarazione agli uffici di polizia. Ho ascoltato l'intervento del Ministro in merito a questi obblighi e le difficoltà che ha esposto per il turismo in Italia.

ma soltanto l'obbligo di denunziare la propria presenza (di dichiarare, cioè, ad un ufficio di polizia la propria presenza), secondo le modalità che stabilisce il Ministero. Credo che ciò sia

al Regolamento in ordine alla nostra discussione. Il nostro Regolamento prevede che il Governo possa presentare emendamenti in qualunque momento ed è il caso che si è verificato oggi: il Governo ha presentato una serie di emendamenti. Siamo nella fase dell'illustrazione degli emendamenti e, poco fa, con molto garbo (il garbo che lo caratterizza), il senatore Nitto Palma ha chiesto chiarimenti al Governo in merito all'emendamento 1.305.

inerente alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. Le offerte pervenute sono state oggetto di verifica da parte della commissione giudicatrice nominata dalla CONSIP. Alcune offerte sono apparse anormalmente basse, ma queste tendevano a far risparmiare alla pubblica amministrazione ben 10 milioni di euro. Quelle strutture, tra le quali la «Qui! Ticket Service», di fatto fornivano agli imprenditori servizi aggiuntivi, che gli stessi imprenditori che ricevono i buoni pasto sono ben lieti di pagare per evitare tempi burocratici e amministrativi eccessivi che mal sì coniugano con la celerità del servizio e il ritardo di eventuali pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Signor Presidente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è intervenuta sulla questione dando ragione ai ricorrenti, ribadendo che se non si ammettessero i servizi aggiuntivi come strettamente connessi con la prestazione in gara si precluderebbe ogni possibilità di sostanziale diversificazione economica tra le offerte e di sviluppare una concorrenza sulla base di una combinazione di fattori dovuta ad abilità imprenditoriali. Questa posizione prende spunto anche da una sentenza del TAR del Lazio in una procedura che ha visto coinvolta proprio la CONSIP. Tali sono i motivi che ci inducono a chiedere ai Ministri competenti un'indagine interna alla CONSIP sulle gare e sulle aggiudicazioni, che nel caso in questione hanno privilegiato multinazionali straniere. Ecco perché è utile, in conclusione, far riferimento a quanto si legge sul sito della CONSIP alla voce «codice etico» nel perseguimento della sua missione la società ha improntato la propria attività ai valori della realtà e dell'imparzialità, della correttezza e della trasparenza; un vero e proprio codice deontologico. Bene, signor Presidente, mi auguro che sulla questione posta dagli interroganti

infatti impossibile orientarsi e soprattutto vi è contraddizione tra alcuni pareri contrari e la successione nella quale saranno posti ai voti gli emendamenti, compresi quelli del Governo, sui quali invece

perché poi ci si possa orientare, di volta in volta, su ogni singolo emendamento, proprio alla luce del parere espresso poco fa. Signor Presidente, non le sembri ingenuo il mio intervento, e mi rivolgo proprio a lei che presiede in questo scorcio finale di seduta l'Aula.

i temi in discussione ci portano ad un dibattito a volte aspro e fatto anche di contrapposizioni. Tuttavia, voglio chiederle (poiché è lei in questo momento a presiedere l'Aula del Senato,

di una dichiarazione fatta da un esponente istituzionale, da un esponente politico, che evoca la rappresaglia come strumento per la soluzione di un qualsiasi problema ed anzi una rappresaglia da uno a dieci. Non ci spaventano parole - come dice il senatore Castelli - sopra le righe, ma credo sia istituzionalmente corretto che lei, che in questo momento presiede il Senato e che è anche il senatore Calderoli, dica una parola di condanna, così la chiudiamo qui e non si lascia un precedente aperto. Senatore Brutti, io non ho espresso un giudizio perché venivano riportate affermazioni fatte in altra sede. Se qualcuno, in questa sede, avesse fatto dichiarazioni del genere in termini di rappresaglia, le avrei censurate come ha fatto lei.